due anni e mezzo, a ventiquattr'ore dalla maturazione di un diritto maturato con i versamenti di due anni e mezzo, dovrebbe decadere, perdendo ogni diritto, sulla base di non so quale considerazione. Ma poiché i giornali hanno dato ampio rilievo (le agenzie ieri e i giornali oggi)

Ma ci sono tanti interrogativi e, se il presidente Grasso li pone, è bene che ce li poniamo tutti. Ci sono molti interrogativi, perché è molto strano - non è un fatto consueto - che ci siano stati ritardi nella proclamazione.

Pertanto, tutti i ritardi accumulati non possono essere scaricati su chi si è trovato, il 13 settembre (ripeto, con ritardi inauditi), non a decidere del destino di un collega ma a mettere la sua faccia su una cosa che non gli piace proprio. Per esempio, a me non piace affatto.

C'è una questione di rapporto tra l'organo Giunta e la Presidenza del Senato. Il collega Giovanardi ha fatto bene a porre la questione, perché noi ci siamo trovati di fronte a due strade. La prima è quella di verificare l'incompatibilità fra l'incarico di sindaco

non c'è alcuna ragione per applicare, nei confronti del collega Cuomo, una tempistica e una procedura diverse. Se la Presidenza del Senato riteneva percorribile invece l'altra strada, aveva tutti i poteri per porre la questione all'attenzione dell'Assemblea e risolverla nei tempi dati.

finestra"). Colleghi, la vicenda in questo momento si chiude qui, perché non è all'ordine del giorno. Capisco benissimo gli interventi che sono stati svolti. Sto svolgendo il ruolo della nuora usata per far sapere alla suocera.

Interverrò in pochi secondi semplicemente per ribadire che, come già detto ieri, la lettera di dimissioni è stata inviata al Senato a fine luglio

fatto benissimo il Presidente a richiamare il senatore Cuomo a fare uno sforzo, perché ne va anche del suo onore.

stato sufficiente che il senatore non facesse alcuna opzione. Così facendo, infatti, il Senato sarebbe dovuto passare alla procedura di decadenza, di cui conosciamo bene i tempi perché - purtroppo - abbiamo avuto due casi di questo genere in questa legislatura. Pertanto, saremmo andati molto, ma molto oltre la fatidica data del 16 settembre.

Dallo stralcio di quell'articolo abbiamo prodotto un nuovo provvedimento, con moltissimo lavoro all'interno della Commissione.

L'esame in sede referente è stato caratterizzato anche da una dialettica molto positiva - lo voglio sottolineare -

Rispetto al testo originario, quello licenziato dalla Commissione ha moltissime integrazioni in risposta a un settore che attende una riforma organica da più di trent'anni. Nella metà degli anni Ottanta, con con la legge n. 163 del 1985 il legislatore intervenne con l'istituzione del Fondo unico per lo spettacolo, il cosiddetto FUS, al fine di ricondurre a un quadro unitario il sostegno statale a diversi settori dello spettacolo, disciplinato da specifiche e numerose

proprio perché tutti sostanzialmente all'interno della Commissione - ma sono sicura anche qui in Assemblea - ritengono che la cultura e lo spettacolo siano elementi fondanti nella vita di un popolo, di una civiltà. In questo

In ogni caso, tengo a sottolineare che è proprio in questa legislatura che siamo riusciti a varare una riforma

che punta a salvaguardare i valori e le identità culturali in questa società globale e tecnologica. Si tratta di una valorizzazione particolare di un aspetto che credo non debba mai essere dimenticato nella sua capacità nella sua capacità e potenza di suscitare emozioni. Tutte le arti dello spettacolo, nella loro grande diversità creativa ed espressiva, sono considerate dall'Unione europea cruciali, in quanto rispecchiano la varietà culturale delle diverse tradizioni e delle storie degli Stati membri. Il nostro lavoro in Parlamento ha permesso di inserire esplicitamente la delega al Governo per il codice dello spettacolo - questa, come sapete, nel quadro delle norme costituzionali nazionali ed europee e delle convenzioni internazionali dell'Unesco, definendo la cornice dei principi fondamentali della Repubblica. C'è quindi una prima parte in cui viene dato questo quadro di contesto e, successivamente, ci sono i principi e criteri direttivi. Sono i decreti legislativi delegati, che consentiranno un'ottimizzazione ed una semplificazione degli interventi pubblici di promozione e di sostegno per lo spettacolo, con l'abrogazione di una serie di disposizioni frammentarie e disorganiche, come ho detto, quelle che si sono via via sovrapposte in questi anni, anche con interventi in sede di manovra di bilancio, che hanno potuto introdurre utili strumenti di sostegno, ma al di fuori di una cornice strategica che in futuro invece sarà chiara, trasparente ed equa. Questo è stato lo sforzo che abbiamo fatto. Per assicurare che tutto ciò avvenga realmente, occorre un organismo capace di valutare sistematicamente e puntualmente l'efficacia degli interventi ed indirizzare le politiche del Ministero ed in questa prospettiva abbiamo creato il Consiglio superiore dello spettacolo. Questo è un elemento molto importante e centrale nella legge, una proposta che è stata accolta dal Ministro con molto favore, perché a questo punto abbiamo il Consiglio superiore dello spettacolo, il Consiglio superiore del cinema ed il Consiglio superiore dei beni culturali. Quindi, c'è un'omogeneizzazione ed un'armonia

e rendendolo uniforme anche rispetto al cinema e all'audiovisivo. Sarà composto da figure di rilievo, figure importanti, persone che dovranno essere coinvolte,

quindi di una scelta che favorisce decisioni trasparenti ed efficaci. Vi è un articolo molto complesso, che vi invito a leggere, che parla della costituzione di questo Consiglio superiore che è un organismo cui diamo molto rilievo.

ulteriori contenuti, è molto stringente. Abbiamo scritto molto in questi sette articoli, perché abbiamo voluto indirizzare con forza il Governo in una certa

per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale. Mi pare che in questi giorni in cui si parla tanto di integrazione e di identità, lo spettacolo e la musica possano essere un elemento potentissimo di integrazione per tutti coloro che si trovano nel nostro territorio, per gli stranieri e per coloro che puntiamo ad inserire e che speriamo

collegano le attività di spettacolo alla nuova disciplina del terzo settore. Abbiamo fatto la grande riforma del terzo settore, ed è presente il senatore Lepri che l'ha seguita, e abbiamo votato a favore di questa legge di cui siamo molto orgogliosi. le associazioni, le imprese e gli altri enti dello spettacolo che rispetteranno le ulteriori condizioni poste dai decreti delegati della riforma del terzo settore, sarà possibile per loro rientrare negli incentivi e nelle agevolazioni previste. una armonizzazione di questi aspetti che riteniamo fondamentali. Il comma 2 introduce una definizione generale delle attività di spettacolo che la Repubblica intende promuovere e sostenere, individuandole in quelle svolte in maniera professionale e caratterizzate della compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico in un contesto unico non riproducibile. Questa è la definizione. Se qualcuno chiede la definizione di spettacolo, andate a leggere quella contenuta nella legge perché vi abbiamo ragionato moltissimo prendendo spunto da fonti internazionali

le attività di musica popolare contemporanea di danza classica e contemporanea. Della danza si parlava naturalmente nei regolamenti ministeriali, ma mai se ne era parlato in una legge e noi, invece, le abbiamo conferito anche questa "cittadinanza" importantissima che fino ad sono le attività circensi perché, come sapete, esiste anche il circo e lo spettacolo viaggiante, le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare perché se facciamo una legge adesso nel 2017 è evidente che dobbiamo pensare anche alle nuove forme di spettacolo.

storia di quel popolo e di quella comunità e, allo stesso tempo, sono anche una proposta culturale e storica vera anche per i giovani di quelle comunità. Per questi motivi abbiamo voluto valorizzare anche le rievocazioni storiche. Tra l'altro c'è anche un altro provvedimento specifico sulle rievocazioni storiche che è all'esame della Camera e che vorremmo portare avanti. Naturalmente riconosciamo anche la tradizione dei corpi di ballo italiani (vedo il

il ruolo degli artisti di strada e delle attività dei centri di sperimentazione: ci sono molte applicazioni di natura tecnologica, quindi abbiamo riconosciuto anche sperimentazione e ricerca, documentazione e formazione nelle arti dello spettacolo.

valenza molto interessante a livello nazionale e internazionale. Ci sono finanziamenti dell'Unione europea che vanno specificamente in questa direzione, quindi ne abbiamo tenuto conto e lo abbiamo introdotto nel nostro testo.

(e nelle deleghe questo sarà scritto con molta chiarezza) spingere molto per l'internazionalizzazione. Il nostro spettacolo, la nostra cultura e la nostra Italia

punti delicatissimi. Signor Presidente, è un punto che non è mai stato affrontato abbastanza e sappiamo quale sia la situazione dei lavoratori dello spettacolo. Li chiamo così,

a incidere sulla formazione del popolo italiano e dei cittadini. Quindi, bisogna capire che è necessario dare un riconoscimento. Questa è una delega che seguiremo con molta attenzione, perché contiene uno dei punti più delicati della legge. I lavoratori dello spettacolo devono essere finalmente supportati in modo diverso.

Abbiamo deciso, in accordo con il Governo, che finalmente ci sarà una distinzione tra i due fondi per cui nessuno, se avrà qualche problema all'interno delle fondazioni, potrà riferirsi a tutto il FUS,

presidenti di Regione a dover curare le gravi situazioni che all'interno delle fondazioni si sono venute a verificare in questi anni. Noi abbiamo detto che la maggior responsabilità

si fa carico di tutte le questioni delicate. Per superare le criticità finanziarie che le fondazioni lirico-sinfoniche affrontano sin dalla riforma degli enti lirici, avvenuta negli anni Novanta, si prevede una responsabilità del sovrintendente sulla gestione economica delle fondazioni.

dovranno rispettare i nuovi parametri al fine dell'inquadramento come fondazione lirico-sinfonica piuttosto che come teatro lirico-sinfonico (la nota questione del declassamento). Abbiamo dato un anno in più rispetto a quanto previsto

per tutto il mondo dello spettacolo. Anche questa è una innovazione molto richiesta, rispetto alla quale si parla dei teatri di tradizione, di istituzioni concertistico-orchestrali (le ICO), di teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, *festival*, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione senza scopo di lucro che svolgono le loro attività esclusivamente nel settore dello spettacolo. Anche questo, quindi, è un aspetto molto rilevante del nostro provvedimento.

abbiamo qualche altro riferimento rispetto alla fondazione lirico-sinfonica che poi si chiamerà teatro lirico-sinfonico. In conclusione, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge rappresenta un vero segnale di discontinuità nei confronti del passato. È una inversione di tendenza per un investimento - come vedrete e avete già visto - strategico stabile sullo spettacolo per valorizzare le punte straordinarie di eccellenza della tradizione italiana e porre le basi per favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro Paese, anche attraverso la cultura e lo spettacolo dal vivo. Chiedo

diffusione della cultura, dell'arte dello spettacolo e anche sviluppo economico. Lo spettacolo dal vivo ha da sempre rappresentato una parte rilevante della cultura italiana e affonda le sue radici in una tradizione millenaria. Il nostro ricco mondo culturale necessitava da ormai troppo tempo di una riforma delle complesse disposizioni legislative in materia di organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche. delle complesse disposizioni legislative in materia di organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche. Andava rivista e razionalizzata la vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, innovando le disposizioni legislative attraverso la redazione di un unico testo normativo denominato codice dello spettacolo. Il codice dello spettacolo, infatti, razionalizza e semplifica procedure amministrative, razionalizza la spesa e incentiva a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, nonché della fruizione da parte della collettività. Il mondo dello spettacolo dal vivo era dunque in sofferenza per la mancanza di adeguate norme, di adeguate risorse, di adeguata e lungimirante visione prospettica, europea e internazionale. Oggi siamo davanti - come ha osservato nella sua relazione la senatrice Di Giorgi - a una riforma organica. Nei mesi scorsi le numerose audizioni della 7a Commissione hanno portato alla luce problemi, limiti e difficoltà dei lavoratori dello spettacolo. Molte sono state le testimonianze di organismi, gruppi di professionisti e associazioni

indispensabili allo sviluppo della nostra cultura e alla coesione della nostra identità, alla diffusione e promozione europea e internazionale della nostra arte, veicolo della nostra offerta turistica. Lo spettacolo dal vivo è però anche occasione formativa fondamentale e - come detto poc'anzi - di contrasto a situazioni di disagio psicologico e sociale,

Non a caso si prevede che le attività dello spettacolo siano realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia e che una percentuale dei flussi sia destinata alle attività nella scuola; ciò a suggellare il valore educativo, formativo e sociale dello spettacolo, un valore sostenuto con tutti i mezzi.

invece trovare un più elevato riconoscimento. E lo sforzo in tal senso sui vari settori dello spettacolo c'è stato e sarà affrontato nel corso dell'esame della delega sul lavoro. Alcuni problemi evidenziati dalle associazioni hanno messo in luce le criticità del sistema previdenziale. In particolare, i musicisti hanno invocato provvedimenti per superare le criticità di alcune normative complesse che determinano il conseguente sommerso; le normative previdenziali; gli eccessivi costi delle tariffe Siae e gli insuperabili problemi economici delle scuole di musica. Finalmente, con il presente provvedimento, potremo dare alle professionalità artistiche dei teatri, della danza, della musica, delle attività liriche, concertistiche e corali, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, dei carnevali storici, delle rievocazioni storiche, ma anche dei complessi bandistici, degli artisti di strada, teatro per i ragazzi, e di tanti altri apporti, degli strumenti importanti di sostegno pubblico e di sviluppo che valorizzino la qualità

all'estero, con un'attenzione a tutti, ma specificamente ai giovani artisti, come già sottolineato dalla relatrice. Finalmente sarà favorito il ricambio generazionale in modo da valorizzare i nuovi talenti e l'attenzione alle nuove tecnologie. La redazione di un testo normativo, il codice dello spettacolo, darà quindi maggiore efficacia e organicità sia alle procedure amministrative, sia alla qualità artistico-culturale

È importante che gli interventi vengano armonizzati con quelli degli enti locali, attraverso accordi di programma. Mi piace infine sottolineare quanto questo percorso legislativo complesso, accuratamente seguito dalla Commissione e accuratamente relazionato relazionato dalla relatrice, sia stato attento alla valorizzazione dell'enorme patrimonio del nostro spettacolo, alle opere dei giovani artisti emergenti, grazie anche a spazi dedicati nelle piattaforme televisive e alla produzione delle nostre opere in Europa e nel mondo. I giovani artisti in particolare, ma pure gli altri lavoratori del settore, potranno accedere a misure di facilitazione attraverso strumenti di credito agevolato. Quanto ai criteri di riparto del Fondo unico per lo spettacolo, sottolineo la centralità dell'erogazione di contributi che valorizzino la qualità delle produzioni e, quindi, finanziamenti in questo senso selettivi a progetti disposti dai giovani di età inferiore ai Non voglio ripetere quello che è già stato detto, ma farò solo un cenno al riequilibrio territoriale: le Regioni colpite dal sisma potranno avvalersi di importanti finanziamenti. Il Consiglio superiore dello spettacolo, infine, ha lo scopo di assicurare compiti di supporto e proposte proposte politiche del settore, di assicurare analisi, monitoraggio e valutazioni alle politiche pubbliche della materia. Concludo esprimendo una soddisfazione viva per la realizzazione di un importante risultato, che vedrà l'aumento delle risorse del FUS, l'instaurarsi di forti collaborazioni con il mondo della scuola, l'estensione dell'*art bonus* a tutto il mondo dello spettacolo, il riconoscimento giuridico a tante manifestazioni che prima non erano riconosciute. La qualità del provvedimento è davvero un grande e responsabile investimento che ci assumiamo nei confronti delle generazioni future. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la discussione di questo disegno di legge, anche in considerazione del fatto che la relatrice ha fatto un'ampia ed efficacissima presentazione di tutte le misure, è un'occasione utile per svolgere alcune riflessioni di carattere generale, poiché contiene una serie di valenze in ambito sociale e lavorativo che vanno ben oltre le finalità esplicite del testo che stiamo esaminando. Viviamo in un'epoca in cui la produzione di beni e materiali di consumo è sempre più legata alle intelligenze artificiali e agli sviluppi delle tecnologie, con la conseguenza di relegare ai margini quelle doti umane che con queste entrano in competizione. In questa ottica la creatività individuale e le capacità artistiche, che trovano forme e modalità d'espressione attraverso attività come quelle teatrali, liriche, musicali o circensi (che sono affrontate in questo provvedimento), acquisiscono particolare importanza, perché contrappongono allo sterile e metallico meccanismo di un processo standardizzato e automatizzato, che ormai non sa più cosa farsene dell'uomo, le dinamiche interattive e situazionali che contraddistinguono le relazioni umane e dalle quali l'uomo, essere sociale per definizione, non può prescindere. C'è la tendenza di considerare le attività culturali come un'attività di svago, come quel lusso in più che ci possiamo permettere se tutto il resto funziona, ovvero quando i conti non sono in rosso, quando il dato di disoccupazione non è una minaccia, quando l'economia tira. Ragionando in questo modo, però, ignoriamo le funzioni intrinseche di quelle attività che possiamo tranquillamente e sommariamente definire culturali.

nel rappresentare storie che sono, appunto, rappresentative delle tematiche che le persone vivono ogni giorno in ambito affettivo, sociale e lavorativo. Le attività culturali sono perciò non solo un diletto, ma costituiscono, anzi, facendo da specchio alla società, il collante con cui essa modella la sua identità e lo fa in modo interattivo, cooperativo. Questo atteggiamento è una delle risposte più potenti alle sfide cui ci pone di fronte il nostro futuro. hanno seguito in modo acritico le idee folli di alcuni *leader*, psicopatici al potere, è scattata una risposta istintiva a queste tragedie, caratterizzata da una valorizzazione spasmodica dell'individualismo, passando però da un estremo all'altro. Oggi dobbiamo renderci conto che questo atteggiamento è non solo individualistico, ma anche egoista, a costo del bene comune. E questo deve trovare una sponda in un'accezione collettiva frutto di processi democratici che, però, sono da imparare. si imparano attraverso modelli nuovi che si possono elaborare anche attraverso le attività culturali, appunto. Favorire il benessere della comunità con la consapevolezza che una rinuncia personale comporta un benessere collettivo che poi fa star bene e meglio

Questa interattività è indispensabile come antidoto a un mondo sempre più connesso attraverso un semplice *click* che, paradossalmente, comporta il rischio di isolamento. Infatti, quel *click* può essere fatto nella solitudine della compagnia di un *iPhone* e, allora, perché scomodarsi a uscire di casa e confrontarsi con altri in relazioni umane quando si può risolvere tutto con un *click*, l'acquisto e il gioco *online*? Pensiamo solo a una delle modalità con cui i giovani risolvono i loro conflitti con i coetanei: premono un pulsante; il che, in caso di cyberbullismo, potrebbe essere una strategia vincente, ma tutto sommato è anche importante imparare dal vivo le convivenze. In questo senso, il neologismo «solitudine digitale» traccia molto efficacemente il nuovo fenomeno sociale a cui possiamo porre rimedio e contrastare attraverso l'attività

Mi sia concesso un breve *excursus* su un altro potenziale che possiamo trovare nelle attività culturali *tout court*, che non a caso sono chiamate anche attività espressive, perché danno accesso a ciò che muove le persone nel loro profondo, le emozioni. A volte quest'Assemblea mi sembra un teatro che ci offre pessimi spettacoli. Pensate se i politici del futuro avessero già oggi l'opportunità di scoprire le proprie emozioni, viverle e metterle a confronto in un contesto disinteressato, potendo così ricevere il dono di fungere da modello. Questa è una delle valenze - diciamo nascoste - del provvedimento in esame che mi inducono a dire che la cultura è non un bene di lusso, ma una materia prima di cui in realtà non possiamo fare a meno per plasmare il nostro futuro. In linea generale, occorre rendersi conto e agire di conseguenza anche in ambito scolastico, sull'onda della riforma che ha messo mano ad alcune esigenze strutturali emergenti del nostro sistema, a cominciare dall'importanza delle emozioni anche a livello di apprendimento. È ormai di evidenza scientifica il potere delle emozioni positive per garantire un maggior successo nei processi cognitivi di apprendimento. Tali emozioni vanno scovate, scoperte, espresse e valorizzate anche nella pratica quotidiana delle nostre scuole future. Si tratta di un processo che può essere valorizzato attraverso attività culturali di cui il disegno

studenti. Pensate che la mortificazione, la punizione e anche lo stesso voto che noi ci arroghiamo di dare agli studenti scatenano delle emozioni negative che inibiscono il processo di apprendimento. Al contrario, le emozioni positive come l'apprezzamento come l'apprezzamento e l'incentivazione costituiscono quasi un fertilizzante per quei processi neuronali e neurofisiologici che devono avvenire nel cervello per rendere

Concludo tornando all'argomento che ho introdotto in apertura: l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie che stanno sempre di più sostituendo l'uomo; uno sviluppo che comprensibilmente viene vissuto come una minaccia e che richiede la ridefinizione del tema lavoro. Il disegno di legge in esame va considerato anche in questo senso una risorsa che si prefigge di maggiorare la considerazione sociale del settore che, oltre ai suoi fini - chiamiamoli nobili - di espressione artistica, con tutte le valenze che ho cercato di elencare, è un contributo a una ridefinizione dei lavori del futuro.

poiché sempre più il lavoro viene eroso proprio dalle nuove tecnologie, dobbiamo trovare altri settori che riconosciamo anche a livello sociale,

per il lavoro prezioso che, insieme ai componenti della Commissione, ha svolto in questi mesi complessi di lavoro, che hanno portato il Senato oggi a esaminare - e ci auguriamo ad approvare a breve - un disegno organico che riorganizza le disposizioni in materia di spettacolo dal vivo

è stata ed è una legislatura molto ricca, prolifica in materia di promozione culturale, di intervento culturale, tanto da consentirmi di affermare che, dopo anni di inerzia, finalmente si torna a scommettere sulla cultura come chiave per costruire il futuro. quindi, il rappresentante del Governo e ringrazio il ministro Franceschini. Ritengo che su questo punto, forse, occorre aprire un ragionamento perché la forza del provvedimento e l'energia che Rosa Di Giorgi ha messo nell'illustrarlo solo la conseguenza di un lavoro che stiamo portando da alcuni anni, in particolare nell'attuale legislatura, per rivedere insieme il potenziale straordinario che l'Italia ha, ha, ovvero il patrimonio culturale, le attività culturali, le istituzioni storiche e i giovani talenti. È attraverso diversi provvedimenti che tutto questo viene fuori

sempre a pungolare il Governo e la maggioranza - il bilancio della cultura torna a superare 2 miliardi questo un obiettivo che ci eravamo prefissati e abbiamo raggiunto, e di cui siamo orgogliosi. Questa è la legislatura dell'*art* *bonus*, in cui 4.250 mecenati hanno donato circa il Sottosegretario mi perdonerà se non sono precisa - 158 milioni e hanno finanziato 1.150 interventi.

degli oltre 45 milioni di ingressi nei musei, i 500 euro per i diciottenni, l'integrazione della politica culturale con la politica dell'educazione e della nuova scuola.

costruire il futuro. E, nel merito, questo provvedimento va in quella direzione. Le istituzioni culturali e lo spettacolo dal vivo avevano bisogno di una riorganizzazione di una riforma strutturale. Le leggi di settore, che avevano ovviamente negli anni Ottanta istruito e promosso positivamente determinati settori, venivano sfiancate dalle

quindi, che con le disposizioni in materia di spettacolo dal vivo contenute nel provvedimento in esame entriamo nel cuore di un'area importantissima di sviluppo culturale ed Sono importanti persino i primi articoli, quelli in cui si specifica quali sono gli obiettivi dello Stato e della Repubblica,

perché il riordino dello spettacolo dal vivo non sia un fatto burocratico, ma rientri in una coscienza collettiva del Paese, in cui l'identità nazionale diventa un obiettivo importante e veda

e la delega al Governo è opportuna e necessaria, perché diventano idrovore che assorbono troppe risorse rispetto alle aspettative del territorio.

le fattispecie di spettacolo dal vivo e anche in questo campo ci sono innovazione e volontà di percepire quanto nel territorio, nelle nostre belle città,

Il consiglio superiore dello spettacolo - come ha detto la relatrice - è un organismo nuovo, parallelo ad altri, per cui non vi è disorganicità nei diversi settori ma finalmente un'organicità degli strumenti consultivi che devono essere effettivamente di supporto e oggettivamente quei luoghi in cui si elabora un discorso di identità e promozione nazionale. Inoltre voglio sottolineare - e per questo ringrazio particolarmente la relatrice e naturalmente il Governo che è stato d'accordo

per l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo e misure in favore di attività culturali nei territori colpiti dal terremoto. Questa è la prima volta che in uno strumento non per l'emergenza, e quindi in uno strumento di altra natura, in uno strumento organico sullo spettacolo, si pensa alle aree terremotate e si dice che la ricostruzione non è solo ricostruzione delle case

diventa essenziale per uscire da uno stato di emarginazione, di solitudine e di rincrescimento nei confronti dello Stato che sembra tanto lontano. Ringrazio, quindi, per questo provvedimento perché non ci sarà mai rinascita dei territori se pensiamo solo alle case e

Ma - come si suol dire - qualche volta il diavolo si nasconde nei dettagli e il disegno di legge contiene un dettaglio - che dettaglio purtroppo non è che profila un aspetto che reputo sicuramente incostituzionale, e comunque surreale, senza fondamento, nel momento in cui stabilisce che, in tema di attività circensi, delega il Governo a rivedere le disposizioni in vigore, arrivando alla graduale eliminazione eliminazione - attenzione: eliminazione e non riduzione - dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse. Con il disegno di legge in esame deleghiamo il Governo a mandare a casa migliaia di lavoratori circensi.

avrò modo di leggere nelle sue parti più significative per mettere il luce il rapporto quasi familiare tra i lavoratori del circo e i loro animali,

e naturalmente quando vediamo i cani salvare dalle valanghe o dalle macerie del terremoto persone che hanno bisogno di soccorso, è uno scandalo, perché quegli animali vengono addestrati e fatti lavorare.

ovunque e sempre gli animali vanno trattati in maniera tale da non subire danni, che il benessere animale va in tutti i modi esaltato,

LAV. L'importo pagato dall'allevatore o dal commerciante o da chi in qualche modo lavora con gli animali (ad esempio un ippodromo), lo incassa la LAV.

se queste centinaia di denunce sono infondate paga lo Stato, se sono fondate c'è un risarcimento incassato dalla LAV. Vi rendete conto della perversione di questo sistema?

e un loro collaboratore. Per loro rappresentava un patrimonio importantissimo. Alla fine l'hanno incastrata in un cortile e, malgrado quelli del circo avessero supplicato le guardie e i vigili urbani di non sparare una dormia perché la giraffa ha una fisiologia particolare,

Dobbiamo metterci d'accordo qui in Senato: il palio di Siena lo vogliamo tenere o lo vogliamo abrogare? La Brambilla lo vuole abrogare e io, invece, lo voglio mantenere. Facciamo un dibattito su Siena e su altre manifestazioni

Capisco benissimo che le persone oggi trovino negli animali una fonte di compagnia e di

a che titolo chi contesta la presenza degli animali nei circhi tiene un animale di quella stazza in un appartamento. Bisognerebbe dire che chi vuole un animale deve avere un cortile o un giardino o, addirittura, dovrebbe farlo vivere in una situazione di libertà perché essere costretto all'interno di un appartamento, magari anche vestito o svestito in estate secondo la moda, può essere una violenza sugli animali. però, non arrivo a quelle conclusioni, ma a conclusioni totalmente diverse e, cioè, che una volta che l'ordinamento giustamente si preoccupa del benessere degli una volta che ci sono norme specifiche perché a tutti i livelli venga mantenuto il benessere animale,

si sarebbe fatta marcia indietro. Siamo in infrazione europea e l'Europa ci ha detto che non potevamo farlo. Però dopo quattro anni la frittata è stata fatta e i topi sono salvi.

con un tavolo di animalisti che è finita con l'auspicio di una signora che il senatore Giovanardi finisse in un forno crematorio, perché contestavo il fatto che le zanzare che portano la malaria dovessero essere debellate.

a Roma abbiamo questa recrudescenza di infezioni, signori animalisti, estremisti talebani,

migliaia di persone nate senza arti in situazioni drammatiche perché non avevano sperimentato sugli animali e sulla cavie incinte. Se lo avessero fatto, ci saremmo risparmiati migliaia di migliaia di persone che hanno passato la vita in una situazione a dir poco drammatica. Nel momento in cui si va nella logica della proibizione, si va in una logica surreale. Quanto al mondo dei circhi e dello spettacolo, cercato con il Ministro - devo darne atto anche alla relatrice - di aver fatto tutto il possibile per fare una cosa ragionevole. Qualcuno mi deve spiegare che senso ha la proibizione: i circhi no, e tutto il resto?

perché ammazzano altri animali, ma se non trovano delle prede, i loro cuccioli muoiono di fame, o li mangia un coccodrillo. La natura è fatta così: è di una cattiveria incredibile. Vogliamo chiudere gli zoo?

Perché nel circo no e nel cinema sì? Perché nel circo no e nella corsa dei cavalli sì? Perché nel circo no e al palio di Siena sì? Perché nel circo no e negli appartamenti delle persone sì?

però gradualmente. La proibizione è totale, ma la graduale proibizione vuol dire che si arriva a proibire totalmente l'uso degli animali magari dando un po' di tempo per eliminarli, cioè per morire: perché è sicuro che, una volta eliminati gli animali, hai ucciso il circo e la sua tradizione, la sua storia, i suoi artisti. Stiamo parlando di spettacoli in linea generale. Nel crollo dello spettacolo, del cinema, del teatro e quant'altro, l'unico settore, anche se gli danno quattro soldi;

faremo cose incredibili, cancellando tutto il nostro passato, andando dietro a talebani, visionari e alle persone che vogliono distruggere tutto. Ma le cose andrebbero motivate. Vi è tutta una serie di emendamenti, presentati dai colleghi della Lega e da me, che chiedono una cosa molto semplice: invece di una graduale eliminazione, una graduale diminuzione.

proibizione? Queste domande le pongo e le riporremo con gli emendamenti. Mi sembra che trasformare l'eliminazione in una riduzione sia una misura ragionevole.

Invito poi qualcuno di quelli che sostengono queste posizioni a presentarsi a Siena, magari il giorno prima del Palio, e andare a fare un dibattito con la cittadinanza senese sul Palio di Siena e sull'utilizzo dei cavalli. Auguri! Si presentino

Quindi, questo provvedimento evidentemente, così come costruito, noi non lo voteremo. Se verrà modificato in questo punto di principio fondamentale, invece, ben volentieri daremo il nostro contributo. PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giro. Ne ha facoltà. Signor Presidente, mi hanno insegnato che in politica bisogna avere soprattutto una qualità: la memoria. Altrimenti il rischio è di fare solo della retorica. Bisogna ricordare i fatti. Si tratta di fatti anche abbastanza banali, banali, che appartengono ormai alla cronaca parlamentare e politica, alle vicende del nostro Paese, che sono fortemente correlate al mondo della cultura. Fortunatamente, infatti, l'Italia è un Paese straordinario dal punto di vista del paesaggio, che è molto diverso e molto ricco, soprattutto per quanto riguarda la cultura. In questa sede ho ascoltato con grande interesse sia la relazione introduttiva della relatrice, sia gli interventi che mi hanno preceduto

completamente modificato il quadro normativo allora vigente, che prevedeva il fondo di garanzia, cioè soldi buttati dalla finestra per film mai fatti, non mai visti. Qualcuno, infatti, potrebbe sostenere che una

Sono stati dati soldi con il fondo di garanzia, il fondo Veltroni, per mille miliardi di lire conteggiate. Vi è un manuale del collega Brunetta molto illuminante, che inviterei a leggere,

con sommessa malizia - stranamente molti di questi registi intellettuali, organici perché fedeli al dettame gramsciano che la cultura è essenzialmente potere, dominio politico, quindi

sull'utilizzo di questi mille miliardi di vecchie lire per il cinema italiano mai fatto e mai visto, il cinema del profondo rosso, senza alcun riferimento a Dario Argento.

il minimo garantito, entrando in un campo minato, quello del cinema italiano dominato dalle sinistre unite, unitissime in quel caso, dall'estrema sinistra alla sinistra di Governo.

che naturalmente deve verificare la qualità del prodotto, la sua appetibilità internazionale, il suo collegamento con i mercati; ma quel sistema è un sistema berlusconiano; 2004:

l'hanno definito: hanno scritto dei libri sui barbari al potere; il grande Settis, *guru* della cultura nazionale, che tanti danni ha provocato per questo Paese (e io ne so qualcosa da quando ero sottosegretario ai beni culturali), ci ha definito dei barbari; sempre nel 2004, ma a gennaio, qualche mese prima della legge cinema, i barbari hanno approvato il codice Urbani sul paesaggio e i beni culturali. Cioè la Carta costituzionale, a difesa del patrimonio culturale tutt'ora

italiana, che ha prodotto fino a 300‑350 milioni di debiti. Questa è la realtà: abbiamo fatto il codice dello spettacolo

legge Veltroni, che ha trasformato gli enti lirici di diritto pubblico in fondazioni di diritto privato. È un obbrobrio giuridico, perché non si capisce chi fa cosa, tra Stato, pubblico e privato, e ha prodotto i guasti che conosciamo.

dopo diciassette, diciotto ore di dibattito, proprio perché volevamo confrontarci? Non era una legge delega, ma una legge di sistema. Noi quella legge l'abbiamo voluta, come dice Bondi, per salvare la lirica italiana, perché all'epoca,

doveroso introdurre criteri di trasparenza amministrativa. Soprattutto abbiamo chiesto ai sindacati di ridurre la parte dei contratti integrativi aziendali e di tornare al contratto nazionale, che non si faceva da decenni, e che era stato rimpolpato con una serie di contratti integrativi che avevano disseminato privilegi ovunque. Ebbene, si sono sollevati gli scudi dei sindacati e, allora, nel 2010, la sinistra si è schierata a difesa del sindacato corporativo. Noi abbiamo tenuto botta, ma il provvedimento è stato depotenziato; eravamo al Governo, non abbiamo chiesto la fiducia, abbiamo trattato con la sinistra portavoce dei sindacati

poste nuove, capitoli di spesa, criteri mai applicati. Adesso abbiamo la legge delega. Questa legislatura sarà ricordata per i voti di fiducia e le leggi delega.

stanze del Collegio Romano. Questo è inaccettabile.

che riguardano la cultura, lo spettacolo, ma anche l'economia del nostro Paese sotto molti punti di vista. Vi è incertezza su quelli che saranno i futuri provvedimenti che adotterà il Governo rispetto a pochi articoli in cui sono elencate alcune intenzioni e alcuni obiettivi, che dovranno evidentemente trovare sostanza attraverso l'azione del Governo stesso. Non possiamo perciò dare una piena e totale fiducia

Vorrei toccare un punto che è stato oggetto dell'intervento del collega che mi ha preceduto: il futuro delle fondazioni lirico-sinfoniche. Sono alquanto preoccupato per l'atteggiamento che sta emergendo in Assemblea rispetto a tali istituti.

(FUS) tra quelle che verranno destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche e quelle che verranno, invece, destinate a tutti gli altri settori della cultura italiana, dal teatro alla musica, alla danza, agli spettacoli viaggianti, ai carnevali e alle rievocazioni storiche, che vengono aggiunte alle discipline che possono essere oggetto della distribuzione di tali fondi. Ho colto in questa affermazione una sostanziale posizione entusiastica e favorevole e una certa rigidità rispetto alle risorse che verranno destinate alle fondazioni liriche.

Sono state definite da una collega del Partito Democratico delle "idrovore"; anche questa è una connotazione molto negativa. Chi mi ha preceduto ha avuto un atteggiamento sostanzialmente analogo, affermando che le fondazioni assorbono tante risorse che vengono gestite male. Io vorrei però mettere in evidenza anche la situazione di alcune fondazioni, che invece producono non solo cultura,

Vengo da quel territorio e conosco la storia di questa gloriosa Fondazione, che ha più di cento anni di storia, in quanto i primi spettacoli lirico-sinfonici e il primo festival risalgono al 1913. Ha una grande storia ha un'importanza fondamentale per il territorio non solo veronese, ma dell'intero Veneto. Vorrei ricordare che il turismo rappresenta una delle poche industrie che producono ancora reddito e che sono ancora competitive in Italia, sulla quale dobbiamo assolutamente continuare ad investire. Quindi i fondi stanziati

della Fondazione Arena che si è recato durante la stagione estiva ad assistere al festival areniano è arrivato a 380.000 unità, cioè 380.000 persone che si sono recate

non solo culturale, ma è un patrimonio turistico-imprenditoriale che noi dobbiamo tutelare; e non possiamo seguire la moda affermando che, siccome rappresentano dei costi per le casse dello Stato, vanno in qualche modo ridimensionate. noi abbiamo corso il rischio di una liquidazione coatta della Fondazione Arena: un rischio dovuto sicuramente ad alcune inadempienze nella gestione; questo è C'è stato un intervento del Governo che, attraverso il commissariamento, ha cercato di mettere in ordine le cose, con un operato virtuoso dei commissari individuati dal Ministro. Ci tengo anche dire che noi, come forza politica, abbiamo sollecitato l'individuazione del commissario, quindi non siamo stati ostili a questa soluzione, perché evidentemente era necessaria. Però vorrei ricordare anche che se la Fondazione Arena e credo anche tutte le altre sono in difficoltà è perché in questi anni sono stati operati tagli consistenti agli enti locali. locali. Le fondazioni non hanno vissuto in questi anni solo dei contributi statali (del FUS), ma hanno vissuto anche dei contributi degli enti locali; mi riferisco alle Regioni, ai Comuni, alle Province e alle camere di commercio. Ebbene, è evidente che con l'atteggiamento degli ultimi Governi di rapina delle risorse degli enti locali, sono venuti meno anche questi contributi. La Regione non può più dare risorse adeguate, non lo può fare il Comune e non lo possono fare le camere di commercio, per la riforma che avete attuato e che ha ridotto diritti camerali, quindi le risorse da reinvestire sul territorio. Quindi, al di là delle risorse del FUS, più o meno omogenee negli anni, c'è stata una scelta dello Stato centrale di penalizzare i territori e gli enti locali, con ricadute anche sulle realtà turistiche e e culturali, che vivevano di questi contributi. Pertanto, c'è una responsabilità ben più ampia dello Stato nella crisi delle fondazioni, che quindi non è esclusiva di chi le ha gestite. Serve il contributo dei privati, anche nella gestione delle fondazioni? Sicuramente sì, l'*art bonus* è stata una scelta positiva. Vorrei però mettere in evidenza che

compenso e anche la riduzione di due mesi dell'attività lavorativa durante la stagione invernale. Ci sono quindi stati degli sforzi che devono essere riconosciuti e apprezzati e non devono essere sviliti da un atteggiamento ostile da parte del Parlamento, né tanto meno del Governo. C'è stata la possibilità di aderire alla cosiddetta legge Bray e da questo punto di vista vorrei sollecitare il Governo a stanziare quei fondi

La Fondazione Arena di Verona ha onorato gli impegni e ora spetta al Governo, attraverso i fondi previsti nella cosiddetta legge Brey, dare quella liquidità che è fondamentale per la sopravvivenza di questa prestigiosa istituzione.

di una parte considerata marginale da parte di molti parlamentari, che riguarda uno dei tanti settori dello spettacolo,

la scelta di inserire nel provvedimento in esame una norma che introduce come obiettivi del Governo la graduale eliminazione - non riduzione, come è stato già sottolineato dal

non può essere superato un confine che noi riteniamo invalicabile, stabilendo che, in assoluto e in nessuna circostanza, ci può essere un rapporto essere un rapporto non di sfruttamento, come qualcuno vuole mettere in evidenza, ma affettivo tra uomo e animale, come si manifesta negli spettacoli del circo. Non riteniamo che il rapporto tra uomo e animale all'interno dei circhi sia di sfruttamento

decreterà la morte dei circhi italiani, con la perdita di numerosi posti di lavoro, o, in alternativa, la fuga all'estero di tutte le attività circensi. I nostri circhi lasceranno il nostro territorio in cerca di territori più ospitali che non hanno questa visione ideologica. Mi auguro che in Parlamento, in questa seduta e nelle prossime, si possa avere un atteggiamento più equilibrato e responsabile, capire che la parola «eliminazione» deve essere soppressa; si può rivedere con «riduzione», non è la soluzione ideale ma può essere già un miglioramento del testo. Si può stabilire anche un criterio secondo il quale alcuni animali possono essere gradualmente eliminati mentre altri devono rimanere, perché fanno parte della storia del circo del circo e di questo tipo di spettacolo che noi vogliamo assolutamente tutelare. Ci sono, cioè, i margini per migliorare il testo. Mi auguro che all'interno di questa Assemblea, a differenza di quanto avvenuto in Commissione, ci sia un atteggiamento più equilibrato e responsabile che abbia a cuore anche questo settore della nostra cultura e - perché no? - della

tenuta di tutti i comparti dello spettacolo e della cultura, ma avrà anche ricadute sul mondo del lavoro. Dobbiamo essere assolutamente consci di questo; dobbiamo tutelare chi fa spettacolo, chi fa cultura, ma anche chi porta avanti professioni, magari di nicchia, che magari riguardano poche migliaia di persone, ma che comunque vanno tutelate e rispettate. Questi, a nostro avviso, sono due dei punti deboli di questo provvedimento e ci auguriamo che nell'azione emendativa possano essere corretti e migliorati. Auspichiamo altresì che questa legge delega trovi attuazione da parte del Governo rispettando il ruolo del Parlamento. È una delega eccessiva non solo nei confronti del Governo ma del Ministro, che noi non condividiamo. È una strada che avremmo preferito fosse stata percorsa con un maggiore coinvolgimento delle Aule parlamentari, ma sappiamo che viviamo in una fase di democrazia limitata, ridotta, in cui il Parlamento rischia di assumere esclusivamente il ruolo di ratificatore delle decisioni prese da altri. Noi non ci rassegniamo a questa idea di democrazia. Riteniamo che il Parlamento rappresenti più del Governo i cittadini (il Governo nato nelle Aule parlamentari) e quindi chiediamo un maggiore coinvolgimento su questo provvedimento e in generale sull'azione legislativa da parte del Senato e della Camera dei deputati. *(Applausi dal Gruppo* *LN-Aut)*. PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granaiola. Ne ha facoltà. *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, colleghi senatori, approda oggi in Aula, dopo un lungo lavoro, il cosiddetto collegato spettacolo dal vivo, stralciato l'anno scorso dalla parte sul cinema, che invece è diventata legge e di cui si attende l'attuazione, mediante l'adozione dei decreti dei decreti legislativi, che a loro volta saranno trasmessi per i pareri alle Camere. Rispetto al testo iniziale dell'Atto Senato 2287, quello proposto dalla 7a Commissione presenta significative integrazioni, con l'inserimento degli articoli dal 3 al 7. Il Gruppo MDP dà quindi un giudizio complessivamente positivo del provvedimento, 11,39)** (*Segue* GRANAIOLA). Nell'articolo 1 della legge al nostro esame sono contenuti i principi sullo spettacolo dal vivo, sui quali sarebbe ben difficile dissentire. Qualunque cittadino dovrebbe riconoscersi in tali principi, visto che la loro enunciazione si ancora ai valori della Costituzione, che su questo punto fanno tesoro della grande tradizione culturale italiana nel teatro, nella musica, nella produzione spettacolistica popolare dei territori e nella rievocazione storica. Il comma 1 precisa che la Repubblica promuove e sostiene lo spettacolo come fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale. Si fa riferimento anche al valore educativo e formativo di queste forme di espressione che hanno - è persino banale ricordarlo - profondità storica e tradizione. Il comma 2, oltre a fornire una definizione generale delle attività di spettacolo che la Repubblica intende promuovere e sostenere, elenca anche i settori di attività con alcune integrazioni importanti, come, ad esempio, le attività di musica popolare contemporanea, le attività circensi, di spettacolo viaggiante e soprattutto i carnevali storici che chi, come me, vive in una città dove si svolgono, sa quanta importanza hanno come espressione artistica e ingegneristica e dal punto di vista turistico, data l'enorme affluenza di pubblico che essi procurano. Il comma 4 precisa e promuove le finalità dell'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo, intervento che deve favorire e promuovere, prima di tutto, la qualità dell'offerta artistica, i progetti innovativi, la trasmissione dei saperi e, oltre a tante altre cose, le modalità di collaborazione fra Stato ed enti locali per l'individuazione di spazi ed immobili non utilizzati o di beni confiscati da concedere per le attività di spettacolo. Nella delega legislativa prevista dall'articolo 2, volta al riordino ed alla razionalizzazione del settore, sono previsti i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega, tecnicismi su cui non desidero intrattenere l'Assemblea. Mi riferisco in particolare al comma 4, lettera *e)* nella parte in cui si trattano i criteri di tipo tecnico-matematico per il riparto delle risorse. Da questo punto di vista, spero davvero che questa legge metta fine alle elemosine *ad personam*, come il discutibile versamento

Per il resto, forse, si poteva togliere qualcosa nella delega, che appare molto, forse troppo, ampia e disciplinare direttamente i vari aspetti con la legge. Comunque, nel corso dell'esame in 7a Commissione, che ringrazio per il lavoro svolto, sono state presentate ed accolte alcune proposte emendative e subemendative che hanno seguito tre filoni principali di intervento: la tutela dei lavoratori impiegati nel mondo dello spettacolo, con particolare attenzione agli aspetti retributivi, la promozione della diffusione di opere di giovani artisti e compositori emergenti, la più ampia fruizione dei contenuti dello spettacolo dal vivo da parte delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle Convenzioni internazionali ed applicabili in materia, in linea con quanto previsto anche nella legge

volte a diminuire la disparità territoriale fra Nord e Sud Italia e fra centro e periferie ed assicurare una maggiore offerta di spettacoli destinati ad un pubblico giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni e l'incentivazione di un'adeguata contribuzione

A mio parere, sarebbe stato necessario porre un termine, perché non è l'immaginario collettivo - e mi rivolgo alla relatrice che ci fa chiedere questa eliminazione, ma la constatazione, anche personale ed anche da parte delle associazioni animaliste, che nei circhi troppo spesso gli animali non ricevano il trattamento che dovrebbero ricevere. Una notazione di carattere critico devo farla anche con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, che spesso versano in condizioni non favorevoli e per le quali c'era sicuramente bisogno di maggiori risorse. Penso di frequente ai lavoratori precari del settore musicale, che contribuiscono ad arricchire la vita di tutti noi e che davvero patiscono una situazione gestionale non ottimale. Non possiamo negare che vi sono situazione di cattiva gestione che nessuna legge, di per sé, potrà sanare. Voglio, a questo proposito, ricordare

La conduzione artistica e amministrativa di un ente che deve produrre e diffondere la cultura come i teatri e le arene storiche non è solo questione di norme ma di persone, di onestà, di spessore umano e, per l'appunto, culturale. Noi abbiamo avuto diversi enti commissariati i quali, con la gestione commissariale, si sono rialzati non perché vi fossero norme diverse ma perché si sono introdotte buone pratiche, oculatezza e ragionevolezza nei rapporti di lavoro e negli acquisti. Sotto questo profilo, l'organismo nuovo previsto e disciplinato nell'articolo 3, vale a dire il consiglio superiore, dovrà, nella pratica, essere un ente che davvero dia indirizzi di concretezza e di buone prassi e che spinga il Ministero a fare una vigilanza seria, non poliziesca e burocratica ma di sostanza e di accompagnamento nella verifica del raggiungimento degli scopi scopi degli enti finanziati. Credo che questo consiglio possa davvero svolgere un lavoro molto importante, se però visto nell'ottica di cui ho detto. *(Applausi

*(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, il provvedimento che discutiamo oggi, intitolato «Delega al Governo per il codice dello spettacolo» nasce dallo stralcio dell'articolo 34 del disegno di legge di disciplina del settore del cinema e dell'audiovisivo, e dell'audiovisivo, divenuto legge nell'ottobre del 2016. In questo modo si è voluto creare *ex novo* un disegno di legge per disciplinare appositamente le attività teatrali, liriche, concertistiche, circensi e dello spettacolo viaggiante, tenendolo ben distinto dalle disposizioni riguardanti il settore cinematografico. Si tratta di norme nate nel tentativo di coniugare le funzioni di aggregazione sociale e diffusione culturale che devono essere necessariamente riconosciute allo spettacolo

dal provvedimento, con la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, che viene incrementata, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di 9.500.000 euro e di 22.500.000 euro a decorrere dal 2020. A ciò si aggiunge poi il fatto che, trattandosi di una delega al Governo, l'ennesima di questa legislatura, gli spazi di manovra del Parlamento sono molto limitati. Siamo potuti intervenire solamente sui principi e i criteri di cui l'Esecutivo dovrebbe tenere conto nel momento in cui andrà a definire

Tra queste: l'armonizzazione e il coordinamento degli interventi economici statali con quelli degli altri enti pubblici territoriali; la definizione dello *status* giuridico di artista lirico, figura professionale quasi sempre in balìa del teatro o della fondazione lirica per cui lavora a causa della sua debole forza contrattuale; la valorizzazione delle realtà musicali legate al territorio, nonché di quelle capaci di coniugare nei loro progetti tradizione e innovazione. Continuando con la sintetica esposizione delle proposte emendative, vorrei soffermarmi sulle condizioni dei lavoratori del comparto, soprattutto dei giovani, gli unici probabilmente a garantire una produzione artistica originale e creativa. Giovani che, nonostante siano vittime del precariato e soffrano dell'assenza di ogni minima tutela contrattuale e contributiva senza che venga loro riconosciuto alcun merito, rappresentano comunque la spinta propulsiva e innovativa del settore. Per questo ho proposto il riconoscimento di premi e incentivi per quei teatri che inseriscono nei loro *cast* giovani artisti

volta a riconoscere le prove di spettacolo come periodo lavorativo effettivo con obbligo di retribuzione, nonché una rimodulazione ed estensione degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori dello spettacolo e, più in generale, alla professione artistica. previsione di incentivi, sotto forma di credito d'imposta, per i gestori di sale da concerto che ospitano orchestre giovanili e sale teatrali adibite all'incentivazione della cultura teatrale per i giovani.

e mi auguro che anche il Governo presti la dovuta attenzione quando passeremo al loro esame. Un altro settore al quale abbiamo dato importanza è quello della danza, per il quale ho proposto l'adozione di norme organiche per la promozione delle attività danzanti e per un migliore funzionamento delle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche. In quest'ambito sono stati approvati, oltre ad un ordine del giorno, anche un emendamento che impegna il Governo a estendere anche alle associazioni culturali che promuovono la danza le agevolazioni fiscali attualmente vigenti per le associazioni sportive dilettantistiche;

Si tratta di un risultato importante perché permette a tutte le famiglie che decidono di iscrivere i propri figli a una scuola di danza, di avere maggiori certezze circa la professionalità e l'effettiva preparazione degli insegnanti. non per importanza, passaggio sulle fondazioni lirico-sinfoniche, per le quali nel corso di questa legislatura sono state prodotte numerose disposizioni normative finalizzate a fronteggiare e risolvere una crisi del settore che, invece di imputare banalmente alla presunta mancanza di fondi, sembra si possa concretamente addebitare alla scarsa presenza di pubblico, poco propenso a partecipare a spettacoli riguardanti la tradizione musicale italiana. Si è intervenuti sul riassetto della *governance* delle fondazioni, sui parametri di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), sulla previsione dei piani di risanamento economico-finanziario, ma l'intervento legislativo appare

Riguardo una gestione più oculata ed efficace delle risorse, auspichiamo davvero che ci siano interventi incisivi, che possano produrre seri benefici e non possono esserci se non si affianca un serio piano di educazione musicale in ambito scolastico e quindi l'insegnamento obbligatorio della musica già dalle scuole dell'infanzia. In un Paese come l'Italia, con un patrimonio musicale unico, che tutti ci invidiano, è veramente incomprensibile che la musica sia considerata un insegnamento opzionale e non completamento del percorso formativo. D'altronde appare difficile pretendere una maggiore attenzione su questi temi se pensiamo che il precariato dei docenti musicali continua a essere una piaga dei nostri tempi,

In conclusione, occorre un progetto organico, interconnesso, di ampio respiro, che abbia come obiettivo di breve termine la soluzione dei problemi e come prospettiva irrinunciabile la formazione di un grande e appassionato pubblico musicale. *(Applausi PLI))*. Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, il collega Giro ha richiamato quest'Assemblea e ognuno di noi all'esercizio della memoria. In qualche modo ho cercato di farlo anche io, ascoltando la relazione molto completa e articolata di stamattina. Resta però che, dal punto di vista della memoria, detto e scritto nel titolo. Noi abbiamo creato alla metà degli anni Settanta, in determinate condizioni di necessità e urgenza (ricordo che fu un decreto-legge), il Ministero per i beni culturali e ambientali. Rispetto ad allora andiamo a conferire al Ministro per i beni culturali la delega per la normativa sulle

decreto-legge, a chi gli voleva dare niente di meno che il cinema ubicato al Ministero dello spettacolo, disse: "Per carità, il cinema mai!" ciò perché lo vedeva in contraddizione con il Ministero per i beni, cioè un Ministero della tutela del patrimonio, un Ministero che organizzava la burocrazia dell'Italia democratica le leggi del 1939, le famose leggi di Santi Romano, tutt'altro che appartenenti all'Italia fascista, ma frutto tardivo di un'Italia liberale. Rispetto al Ministero voluto e organizzato da Spadolini, nella nostra storia politica e parlamentare direi che, perlomeno dagli anni Ottanta, vi si contrappone tutt'altro progetto,

nell'organizzazione del Ministero gollista, che diverrà poi quello di Jack Lang. Vi si oppongono non solo i conservatori dei beni culturali, ma anche quel mondo non privo di molti sentimenti antisocialisti, il mondo comunista, che è radicato nella nostra archeologia e, ha rilevato il collega Giro con perfidia, anche nella cinematografia dell'Italia repubblicana. Già. Ma la soluzione che abbiamo dato può essere quella di uno strumento come la delega al Ministro? Si cambiano completamente il volto, la natura e la struttura del Ministero senza dirlo, basandosi sulle prerogative del Ministro. Da questo punto di vista, ho l'impressione che lo strumento della delega sia imperfetto, imperfetto, fin troppo abusato in questa legislatura. Tanto più che l'ottima relazione che abbiamo ascoltato stamattina e che il presidente Marcucci ha guidato nei lavori della Commissione, della quale non faccio parte in questa legislatura, a un certo punto dice si è dovuto espungere una norma del testo iniziale del Governo perché qui non abbiamo preoccupazioni di conflittualità tra Stato e Regioni. Se è un auspicio, l'Assemblea non ha difficoltà ad accoglierlo, ma di che cosa stiamo parlando? Tutto il processo normativo che ha portato nell'area del Collegio Romano persino il controllo politico, nel senso comunista e gramsciano, del CONI e delle federazioni sportive è sempre incentrato sul Ministro invece che sul Ministero. Ecco perché, al di là delle ragioni richiamate dai colleghi dell'opposizione,

risposta chiara - poi la si può condividere o no - dal rappresentante del Governo. Il rappresentante del Governo ha il dovere, soprattutto rispetto alle riserve che sono state avanzate da noi dell'opposizione sullo strumento della di contrapporci le ragioni per le quali si può istituire, al fianco di un consiglio nazionale dei beni culturali che era l'unificazione dei vecchi consigli superiori dello spettacolo. Torniamo all'Italia del Dopoguerra, signor Presidente, quando Carlo Ludovico Ragghianti era il Sottosegretario preposto alla non scolarità quando poi il dibattito - mi ha colpito il richiamo della senatrice Blundo - va sull'organizzazione scolastica della cultura e una norma della delega lo consente. Ma cosa c'entra con questo il nuovo consiglio nazionale dello spettacolo? Dove evidentemente non saranno più criteri tecnico-scientifici, ma Credo di avere esaurito il tempo a mia disposizione e mi scuso per aver abusato dell'attenzione dei colleghi. Quello che mi premeva dire è che, per l'atteggiamento del mio Gruppo, oltre alle considerazioni settoriali, ma significative, fatte dall'amico Carlo Giovanardi, sarà decisiva la risposta del rappresentante del Governo, in modo da non condividere finalmente il destino, lo *Zeitgeist* di questa legislatura: disegno di delega e su esso la fiducia, per citare il collega Giro.

a molti mesi di distanza, il Parlamento, dopo aver approvato la parte riguardante il cinema, si accinge a dare la delega al Governo per la nuova disciplina del mondo dello spettacolo e lo fa in un punto limite, sapendo che l'opera iniziata in questa legislatura verrà conclusa solo in parte. Non spetta a me dire se si poteva fare prima. Ora l'auspicio è che l'attenzione e il cambio di passo che ci sono stati in questi anni sulla funzione sociale, ma anche economica, della cultura vengano mantenuti anche in futuro. Sicuramente va dato atto al nuovo Ministero, guidato da Franceschini, di aver dato una svolta in questa direzione. Il provvedimento è significativo, a cominciare dalla volontà di dotare il mondo dello spettacolo di un codice unico. Ci sono ambiti che da tempo necessitavano di una profonda revisione o comunque di un più solido inquadramento normativo. Penso alle fondazioni lirico-sinfoniche e alla necessità di raggiungere una propria sostenibilità economica attraverso una maggiore attenzione alla produzione artistica, ai riscontri in termini di pubblico e al rapporto col territorio e con il tessuto culturale. È importante che si proceda con la revisione dei criteri per l'erogazione dei contributi, come in verità già è avvenuto a partire dall'ultima assegnazione, grazie a una norma contenuta nella legge di stabilità del 2015. Mi riferisco soprattutto al riconoscimento del valore dello spettacolo come indicato nel primo articolo e che la relatrice Di Giorgi ha ben evidenziato, ma anche all'importanza data alle pratiche amatoriali, alle espressioni artistiche popolari, al valore cioè di quella cultura legata alle tradizioni e alla storia di un territorio

alla necessità di favorire il ricambio generazionale, al puntare sulla crescita in termini qualitativi dell'intero settore. Per me sono dirimenti questi tre punti: educazione alle forme artistiche, ruolo dell'associazionismo, nuove generazioni. Esiste, Esiste, nel nostro Paese, una importante realtà di associazioni, di volontariato appassionato e competente, di bande, cori, filodrammatiche e gruppi teatrali, gruppi storici, carnevaleschi e folkloristici, gruppi coreutici, che svolge una preziosa funzione una preziosa funzione di coesione sociale e di educazione alla musica e alle arti più in generale. Sono decine di migliaia di preziose realtà operanti ovunque e in tutti gli ambiti, che garantiscono un presidio culturale territoriale senza il quale l'Italia sarebbe molto più povera e meno attrattiva. Lo hanno ribadito in Commissione soprattutto i rappresentanti del tavolo permanente ed a loro dobbiamo tutti un grande ringraziamento per l'impegno generoso e qualificato che mettono al servizio delle nostre comunità. Ma c'è anche una generazione creativa ed innovativa che è depositaria di nuovi saperi e conoscenze, che ha competenze importanti, in grado di produrre anche valore economico e occasioni di lavoro qualificato. La cultura, anche nelle sue espressioni più popolari, può costituire un volano economico, a dispetto di chi un tempo sosteneva che con la cultura non si mangia. Come dimostrato in diversi studi, i territori più vivi culturalmente sono anche i territori più dinamici e competitivi dal punto di vista produttivo. Occorre allora valorizzare e dare gambe e respiro a tutte queste esperienze che, nella loro varietà, contribuiscono alla crescita del tessuto sociale ed economico del Paese e delle singole identità territoriali. Purtroppo, credo sia questo l'elemento debole del provvedimento che andiamo ad approvare: uno sbilanciamento verso le forme culturali "alte" e una minore convinzione rispetto a quelle forme che incidono sui territori, che mettono in campo un'offerta per un pubblico che altrimenti non avrebbe altre forme di accesso alla cultura. I benefici fiscali con l'estensione dell'*art bonus* in favore delle istituzioni concertistico-orchestrali, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, sono sicuramente elementi positivi. Come lo sono le norme che garantiscono la qualità dei centri di formazione (mi riferisco in particolare ai necessari requisiti previsti per le scuole di danza) e quelle che semplificano alcuni *iter* burocratici che non hanno alcuna seria giustificazione. Ma pur riconoscendo l'alto valore sociale e formativo del volontariato, troppo poco questa legge delega prevede a loro sostegno. Neppure le misure previste, giustamente, a favore delle realtà sportive. Come se la promozione culturale fosse meno importante per il Paese di quella sportiva. Per questo l'invito che rivolgo al Governo è di rafforzare questi ambiti, soprattutto sul terreno delle risorse loro destinate. Non ricevono più nulla dal FUS e ben poco dagli enti locali. Vivono spesso solo della buona volontà dei loro sostenitori. Dobbiamo dare la giusta centralità a quella cultura che arriva nei luoghi più lontani o difficili, quella che svolge un ruolo prezioso in termini di inclusione sociale, quella che è d'ausilio sul fronte sociosanitario, ad esempio coi disabili, e che è tutt'altro che una cultura di serie b. Lo dobbiamo soprattutto alle centinaia di migliaia di persone appassionate e competenti che dedicano gratuitamente il loro tempo alla comunità e alla sua crescita. E lo fanno creando anche opportunità lavorative per i professionisti: pensiamo che nel solo Trentino le scuole musicali e le bande impiegano oltre 500 maestri di musica, formati dai due conservatori attivi in Trentino. Tutte persone che altrimenti sarebbero destinate a non poter esercitare la loro professione. Anche per questo avevo presentato una proposta, purtroppo non accolta dal Governo, per una parziale detrazione fiscale delle spese sostenute dalle famiglie per corsi di insegnamento musicale, al pari di quelle concesse per le formazione sportiva. La relatrice aveva avanzato una sua proposta, apprezzata da tutti, ma purtroppo anche quella si è dovuta ritirare per mancanza di idonee coperture. Adesso, in Aula, l'abbiamo ripresentata come ordine del giorno, confidando che il Governo confermi almeno l'impegno politico ad intervenire nella prossima finanziaria per introdurre benefici fiscali per la promozione delle attività bandistiche, corali, coreutiche, teatrali e folkloristiche che organizzano momenti di formazione riconosciuta per i bambini e i ragazzi. Allo stesso tempo vi è la necessità, che sollecito da inizio legislatura e che ho ribadito anche nel nostro ordine del giorno, di una revisione della disciplina d'autore in favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale per le iniziative, a scopo benefico, di libera esecuzione dal vivo di brani musicali. Ed ugualmente è necessaria l'eliminazione di un'ulteriore quota di burocrazia, costosa ed eccessiva. Non è possibile, ad esempio, che per eseguire un balletto in piazza, senza palco e senza alcun rischio per la sicurezza, occorra una specifica autorizzazione della polizia amministrativa. Tante altre sono state le richieste del volontariato culturale a cui non si è data ancora risposta: un minimo di finanziamento dal FUS, agevolazioni fiscali anche per chi vuole investire sul volontariato culturale, agevolazioni sulle imposte di bollo che oggi spettano solo alle ONLUS, la riduzione delle aliquote IVA per l'acquisto di strumenti, il riconoscimento come realtà formative, una maggiore elasticità nei rapporti di lavoro intermittenti con i collaboratori tecnici, così come avviene per lo sport. Infine voglio soffermarmi su una situazione che si è verificata quest'anno e che ha avuto dell'incredibile. Mi riferisco al fatto che, per l'anno d'imposta 2016, non è stato possibile, non si sa se per dimenticanza o per volontà politica, riservare il 2 per mille dell'IRPEF alle associazioni culturali. Questo, come è facilmente comprensibile, ha messo in difficoltà moltissime realtà che erano convinte di poter accedere a questo tipo di sostegno. La richiesta, contenuta in un nostro ordine del giorno, condiviso dall'intera Commissione, è che nella prossima legge di bilancio questa doverosa misura possa essere reintrodotta in misura stabile. Voglio, poi, fare un ultimo appello al Governo affinché modifichi finalmente - l'ho chiesto molte volte, senza successo - una norma eccessivamente penalizzante introdotta dal Governo Monti, che vieta di attribuire compensi agli amministratori degli enti collegati allo spettacolo. Come possiamo pensare che il presidente di un centro servizi culturali, che ha la responsabilità della gestione di un bilancio da milioni di euro, debba svolgere questo compito assumendosi in proprio tutte le responsabilità, anche penali, senza percepire alcun compenso? In conclusione, esprimo la soddisfazione del nostro Gruppo per questo attesissimo provvedimento, che mette finalmente ordine nel complesso settore dello spettacolo e che affida al Governo una delega molto articolata ed impegnativa. Ringrazio la Commissione cultura e la relatrice Di Giorgi, con cui abbiamo lavorato in un clima costruttivo, e li ringrazio anche per aver tenuto conto nella delega della specificità della realtà culturale della nostra Regione. La sfida è strategica per l'Italia ma anche per i suoi territori, perché gli effetti, dal punto di vista sociale ed economico, per il valore aggiunto che la cultura e lo spettacolo possono e devono dare, sono assolutamente significativi. L'ultimo scorcio di legislatura è un tempo utile per farlo.

colleghi, ricostruendo brevemente le vicende procedurali di questo disegno di legge, ricordo un aspetto significativo. La delega al Governo per il codice dello spettacolo deriva dallo stralcio di una norma originariamente contenuta nella disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo, che poi è diventata la legge n. 220 del 14 novembre 2016. Il disegno di legge oggi in esame ha comunque mantenuto, ai fini dell'esame in 7a Commissione e in Assemblea, la natura di collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016. E ciò è significativo perché dimostra che si è voluto dare maggiore importanza allo spettacolo dal vivo, che avrebbe corso il rischio di essere annacquato all'interno di un provvedimento di rilievo

rispetto alla versione originaria derivante dallo stralcio. Inoltre, ritengo quanto mai fondamentale convergere verso una convinta prosecuzione dell'esame di questa disciplina presso la Camera dei deputati, dal momento che, allo stato attuale, ci troviamo ancora alla prima lettura da parte di questo ramo del Parlamento. Ricordo, a tale proposito, come il Ministero dei beni e delle attività culturali abbia da subito posto costante attenzione e specifico impegno al fine di compiere un esame approfondito e portare a conclusione la valutazione di questa normativa non più rinviabile. Ricordo, infatti, che con la legge 30 aprile 1985, n. 163, il legislatore interveniva in materia con l'istituzione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), allo scopo di ricondurre a un quadro unitario il sostegno statale ai diversi settori dello spettacolo disciplinato da specifiche leggi tra cui, per citare le più importanti, la legge 4 novembre 1965, n. 1213, sulla cinematografia e la legge 14 agosto 1967, n. 800, sugli enti lirici e le attività musicali. A questo intervento sarebbe dovuta seguire una riforma organica dei diversi settori, prevista dalle stesse disposizioni transitorie dettate dall'articolo 13 che testualmente stabiliva: «Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi». Tale riforma, purtroppo, nonostante sia stata annunciata più di trent'anni fa, non è ancora stata portata a compimento. In questa legislatura siamo riusciti a riformare il settore del cinema. Un passaggio fondamentale ma parziale: la disciplina delle attività di spettacolo ha richiesto approfondimenti che sono stati effettuati, ma adesso occorre uno sforzo finale per completare il quadro con l'approvazione della parte del disegno di legge stralciata che disciplina lo spettacolo. Dal punto di vista del merito del provvedimento, il disegno di legge si compone di sette articoli. L'articolo 1, nell'elencare i settori di attività di spettacolo oggetto del provvedimento, specifica che saranno ricomprese le attività teatrali, liriche, concertistiche e corali, ma anche le attività di musica popolare contemporanea, di danza classica e contemporanea, le attività circensi e di spettacolo viaggiante, oltre alle attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare, i carnevali storici e le rievocazioni storiche. Non manca neppure il riconoscimento del valore delle pratiche artistiche amatoriali, delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore, del teatro di figura, della tradizione dei corpi di ballo italiani, degli artisti di strada e dei centri di formazione, sperimentazione e ricerca nelle arti dello spettacolo. Si esplicita che la promozione e il sostegno allo spettacolo si basa sulla considerazione che esso rappresenta un fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, e costituisce anche un valore formativo ed educativo. Le azioni di promozione e sostegno di cui lo Stato si farà carico saranno finalizzate, tra gli altri obiettivi, a migliorare la qualità e la pluralità dell'offerta artistica; ad aumentare le competenze artistiche e tecniche; al coinvolgimento dei giovani attraverso la trasmissione delle competenze, la formazione professionale e il ricambio generazionale; alla diffusione dell'offerta dello spettacolo in maniera omogenea sul territorio nazionale e alla promozione delle iniziative all'estero. L'articolo 2 si occupa delle deleghe al Governo da adottare entro dodici mesi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni che disciplinano le fondazioni lirico-sinfoniche. Ma anche per la riforma dei settori di teatro, musica, danza, spettacoli viaggianti, attività circensi, carnevali storici e rievocazioni storiche, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato "codice dello spettacolo". Tra i principi da seguire nell'ambito della delega, il più importante riguarda la gestione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Le modalità con cui si provvede ai criteri di riparto del FUS e all'erogazione delle risorse - spiega il provvedimento vengono stabilite attraverso decreti da emanare, sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo previa intesa con la Conferenza unificata. Tra le linee guida rientrano, in particolare, la necessità di assicurare la collaborazione dei diversi livelli di Governo e l'armonizzazione degli interventi tra Stato ed enti territoriali anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma, la promozione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti. In questa grande opera di diffusione e promozione rientreranno anche le scuole e gli istituti di alta formazione e l'utilizzo di strumenti di accesso al credito agevolato, anche attraverso convenzioni con il sistema bancario. Per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, il testo approvato dalla Commissione tiene conto degli interventi legislativi adottati d'urgenza a giugno del 2016 che hanno accompagnato l'erogazione di risorse aggiuntive milioni a sostegno delle fondazioni stesse, poi garantite dalla legge di bilancio 2017. Nello specifico, viene previsto lo scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo delle risorse destinate alle fondazioni e il riordino dei criteri di finanziamento con i principi di riparto previsti dalla finanziaria di quest'anno (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019). Si dovrà tenere conto della regola che impone di erogare risorse assicurando prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei contributi provenienti da soggetti privati, Regioni ed enti locali. L'assetto organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche dovrà garantire pratiche gestionali efficaci e idonee a garantire il funzionamento secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità. Il quadro si completa con le disposizioni finali stabilite nell'articolo 7, che spostano al 31 dicembre 2019 il termine per consentire alle fondazioni di adeguarsi ai nuovi parametri, creando di fatto i presupposti per una riforma organica che interessa tutte le fondazioni, non solo quelle in crisi, e favorendo il concorso per il sostegno di tutti i soggetti (Stato, Regioni, enti locali e finanziatori privati). Per i settori di teatro, musica, danza, spettacoli viaggianti, attività circensi, carnevali storici e rievocazioni storiche, il Governo dovrà tenere conto dell'ottimizzazione dei diversi settori, basandosi sui principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti. Il fine è soprattutto di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete e riconoscendo il ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo. Nella definizione delle misure di sostegno dello Stato, i decreti legislativi dovranno introdurre regole per assicurare il riparto sulla base di una serie di criteri che vanno dell'esame comparativo dei programmi di attività pluriennale, alla valorizzazione della qualità delle produzioni.

Si dovrà tenere conto poi dell'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale, del finanziamento di progetti predisposti da giovani *under* 35, dell'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero. Infine, dell'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione, e l'aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo con particolare attenzione a quelli ubicati nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il provvedimento tocca anche la delicata tematica del rapporto di lavoro che, in ossequio all'articolo 36 della Costituzione, deve assicurare ai lavoratori dignità nella retribuzione e nelle tutele: le norme devono disciplinare in modo sistematico e unitario il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, tenuto conto delle specificità e del carattere intermittente delle prestazioni lavorative e delle tutele previdenziali e assicurative. L'articolo 5 prevede due nuove misure a sostegno del settore: l'estensione dell'Art Bonus a tutti i settori dello spettacolo (cioè anche alle istituzioni concertistico-orchestrali,

la misura del credito d'imposta per le opere (prime, seconde e terze) di nuovi talenti; definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. Il beneficio è riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche. In conclusione, l'esame in sede referente ha restituito a quest'Assemblea un provvedimento completo, organico e ricco di novità per il settore dello spettacolo. Con la collaborazione di tutte le forze politiche, la 7a Commissione è riuscita a trasformare una semplice

dei pochi aspetti positivi che contiene il disegno di legge, atteso da tanti anni dai lavoratori del settore, è certamente dovuto all'impegno che la relatrice ha profuso nei lavori della Commissione.

mio avviso, il diavolo si nasconde nell'impostazione generale di un provvedimento che impatta nel settore della cultura, che dovrebbe essere un pilastro della rinascita, anche economica, del nostro Paese.

Vi è anche un po' il pensiero pervasivo che sostanzialmente il settore privato debba intervenire laddove i tagli del pubblico non garantiscano più il funzionamento del sistema. Questo avviene in settori dove invece il pubblico deve avere un ruolo assolutamente

Vorrei iniziare dalla questione dell'accentramento dei poteri. C'è anzitutto una grande questione costituzionale in questo disegno di legge, che non è quella sollevata dal senatore Giovanardi (ancora una volta dissento dal suo intervento).

che sarebbe prima o poi passata una riforma costituzionale che, come sappiamo bene, attraverso le modifiche dell'articolo 117 della Costituzione accentrava i poteri nello Stato centrale. Ovviamente sappiamo tutti com'è finita.

alla questione costituzionale nell'articolo 6, dove c'è una sorta di clausola di salvaguardia che dice che le disposizioni di questo disegno di legge sono immediatamente operative anche per le Regioni a Statuto speciale, fatti salvi naturalmente di statuti regionali. Ma questo non garantirà non ci saranno dei ricorsi, perché il disegno di legge non specifica quali siano effettivamente gli ambiti sui quali la competenza statale potrà generare dei decreti che non siano impugnabili. questo tema ricorrerà, a mio parere, una volta emanati i decreti attuativi. La questione dell'accentramento ricorre anche nell'articolo che istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo.

giusto siano in capo a un organo terzo rispetto al Ministero. Ancora una volta, c'è una sorta di confusione che ritorna anche in altri atti amministrativi di questo Governo riguardo gli organi consultivi e propositivi. Credo si debba fare chiarezza. Una cosa è un organo consultivo e propositivo di nomina ministeriale (ossia i superesperti

rappresentativi della comunità, a cui il provvedimento si riferisce (in questo caso, la comunità dei lavoratori dello spettacolo attraverso le loro associazioni, sindacati eccetera). Il Consiglio superiore dello spettacolo ha 15 membri (non 11, come ho letto erroneamente in alcune parti): 11 membri sono di nomina ministeriale, 4 di nomina anch'essa

Signor Presidente, inizierò anch'io ringraziando la relatrice, senatrice Di Giorgi, perché in effetti le va riconosciuto un approccio incentrato sull'ascolto delle istanze provenienti dalle forze di opposizione. Ahimè, purtroppo, merita molti meno ringraziamenti il ministro della cultura Franceschini, che non ha di certo mostrato il medesimo approccio né nei confronti delle opposizioni né, credo, nei confronti della relatrice, che appartiene forza politica. Una mancanza di ascolto che si è poi tradotta nell'atteggiamento dei suoi baldi rappresentanti dell'ufficio legislativo, poiché il ministro Franceschini era talmente interessato a questo provvedimento - come era talmente interessato al provvedimento di

il "privilegio" di essere molto curate. Forse sarebbe stato bene in qualche occasione dimenticarcene, e invece le abbiamo ricordate sin troppo perché evidentemente si vuole portare a termine quel progetto scellerato, che va avanti da anni trasversalmente, con diversi colori di diversi Governi, che a nostro avviso è lo smantellamento del settore per poi farlo rinascere

che ha creato un mostro giuridico, per cui abbiamo istituzioni di natura giuridica privata alle quali, però, è riconosciuto un interesse pubblicistico. Tutto questo ingenera il caos nel quale sono finite queste fondazioni, dovuto, a nostro avviso, per la maggior parte, non solo a questo mostro giuridico, e quindi anche alle conseguenze che ha avuto, ma anche ai tagli,

hanno provveduto a tagliare insistentemente e costantemente i fondi alla cultura, come se la cultura non fosse importante nella vita di un Paese, come se non costituisse una delle fonti principali anche per la nostra produzione industriale, ma non ho tempo di articolare questo ragionamento. Detto questo, una delle ragioni per cui oggi le fondazioni versano in queste condizioni è la malagestione, derivante dal fatto che anche in questo caso si è perpetrata nel tempo la cattiva abitudine di considerare i ruoli apicali, quindi i ruoli di sovrintendente all'interno delle fondazioni, di direttore artistico ma anche di tutti i vari direttori amministrativi, come un come un *parking* per accontentare amici politicamente vicini, anche se questi amici non avevano di certo dimostrato, in occasioni precedenti, di essere bravi nella gestione di queste fondazioni lirico-sinfoniche o anche se queste persone non avevano *curriculum* *vitae* atti a motivare la loro nomina in quelle posizioni.

di sé stesso, compariva una lettera *b)* in cui si riconosceva l'attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente quale unico organo di gestione.

con i relatori dei provvedimenti se poi è ricomparso un riferimento alla responsabilità nella gestione economica delle fondazioni.

non siamo noi in realtà a dire che in questo provvedimento non si è fatto abbastanza e che in Italia, patria della danza, questa rischia di scomparire. È stato il grande ballerino ed interprete Roberto Bolle a dire

Infatti un conto è l'autocelebrazione e un conto è la sostanza. Ricordava correttamente il senatore Giro che sul cinema e sulla cultura si è fatto molto. Ho l'impressione, anzi la certezza, che l'approccio

neanche le persone per bene che hanno voglia di seguire i provvedimenti riescono a farle. Infatti, l'autocelebrazione di cui parlavo prima porta a poco o quasi nulla di concreto e poi vedremo l'aspetto peggiore. Certo ci sono anche degli interventi.

voi, noi non vogliamo regolarizzare quello spreco enorme di denaro pubblico cui si continua ad assistere?

Avete provato a delegare all'uomo solo al comando, quando avevate il *premier* abusivo Matteo Renzi. Oggi cercate di far credere che sia un lavoro di squadra, ma il Parlamento viene esautorato delle proprie volontà, perché di fatto ci chiedete di votare una delega al Governo. E lo farete probabilmente anche sulla legge elettorale. Non avete il coraggio di portare avanti neanche le vostre convinzioni, come quella sciagurata norma sullo *ius soli.*

il senatore a vita maestro Claudio Abbado e la sua frase molto nota: «La cultura è un bene comune primario come l'acqua. I teatri, le biblioteche, i musei e i cinema sono come tanti acquedotti».

fino alla fine del ciclo scolastico delle scuole medie superiori. È, quindi, evidente che, insieme al lavoro che stiamo facendo oggi, stiamo dando una risposta a quei bisogni di di accesso al patrimonio che sappiamo essere fondamentali. I beni culturali e l'esperienza connessa ai linguaggi artistici del corpo e della mente sono in grado di farci superare le barriere di un carcere, di un ospedale o di un quartiere degradato. Le arti performative, infatti, hanno il potere di abbattere i muri, se non sempre quelli reali, certamente quelli relazionali - e molto è stato detto in questa Assemblea da chi mi ha preceduto - e creano benessere anche in condizioni di disagio, ma soprattutto e per tutto l'arco della nostra vita emozionano e ci fanno vedere al di là dell'infinito. Questo ha molto a che fare con la crescita sociale, con la ricerca umanistica e scientifica. Certo, come ci spiega Carlo Rovelli nel saggio «Sette brevi lezioni di fisica», ci vuole tanto impegno e fatica per comprendere l'equazione di Riemann, ma meno di quelli necessari per arrivare a sentire la rarefatta bellezza

di reinventare anche una nostra capacità di sviluppo sociale ed economico. Sappiamo in questo momento - molti lo hanno sottolineato - come l'impresa creativa, anche in Europa tanto sostenuta, sia uno degli elementi fondamentali, un asse di sviluppo al quale dobbiamo rivolgerci. Lo spettacolo, con le sue visioni, le magie e le narrazioni, rende ancora più attraenti i luoghi della cultura e questo è un altro elemento di non poco conto per quanto riguarda un Paese come il nostro che di luoghi della cultura ne ha così tanti. Nella sua visione più alta - e possiamo sempre lavorare perché lo spettacolo sia valutato nella sua qualità - è uno degli elementi fondamentali della nostra civiltà e, quindi, merita di essere conosciuto, salvaguardato e tutelato anche nelle sue tracce materiali, ma valorizzato nelle sua qualità immateriale.

che ha adeguato la normativa italiana alla convenzione Unesco, estendendo salvaguardia e sostegno a cinque ambiti del patrimonio culturale immateriale, tra cui le arti dello spettacolo, le pratiche sociali, riti e feste e l'artigianato tradizionale. Inoltre, con il decreto-legge n. 146 del 2015, per la prima volta, sono state riconosciute la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale come attività rientranti tra i livelli essenziali delle prestazioni, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione. E questo è stato fatto nella corrente legislatura. La strada è ormai tracciata anche dalla ratifica della Convenzione di Faro, che imprime e promuove processi di partecipato riconoscimento dell'eredità materiale e immateriale da parte delle comunità. In questo senso acquista particolare significato l'inserimento delle rievocazioni dei carnevali storici come oggetti di interesse nella norma che stiamo prendendo in esame. legge in discussione, come elaborato in Commissione - anche io ringrazio la relatrice per il lavoro svolto, il presidente Marcucci, il Governo e il Ministro Franceschini, che ha condotto insieme a noi questo lungo percorso ha opportunamente indicato i riferimenti nazionali ed europei ai quali si ispira il nuovo codice dello spettacolo, in manifesta coerenza con il lavoro svolto da Parlamento e Governo in questi anni.

importante a livello di aggregazione sociale e di implementazione della creatività dei giovani,

non abbiamo memoria non solo di quello che è stato fatto, ma nemmeno di quello che stiamo facendo. Ciò perché - mi auguro con un'ulteriore precisazione a livello emendativo in Aula - verrà fatto riferimento al fatto che

dove vediamo lavorare insieme il MIBACT e il MIUR, insieme al terzo settore, e quindi con tutto quel volontariato anche culturale che qui si è citato, per poter mettere veramente a sistema quello che nell'ambito culturale viene fatto, ma che spesso vede poco interfacciarsi i vari mondi formativo e produttivo ed anche i vari livelli di promozione, e quindi il terzo settore, il settore del privato sociale con gli enti pubblici e quant'altro. Noi abbiamo inserito invece queste queste logiche di sistema nei tanti provvedimenti di cui ci stiamo occupando negli ultimi mesi e sui quali continueremo a lavorare. Un punto importante è il *welfare* dei lavoratori dello spettacolo,

euro. Su questo davvero credo che la delega sia stringente e preveda che ci siano poi dei testi specifici.

I momenti della bellezza, dell'aggregazione, della libertà creativa devono restare i baluardi della nostra civiltà e convivenza civile. Le arti, e certamente anche quelle dello spettacolo, sono frutto della libertà creativa individuale e collettiva; quella dimensione aperta al confronto che guarda al futuro elaborando nella contemporaneità quello che il pensiero, anche il più antico, ci mette a disposizione. Questa è la visione estetica ed etica

Carozzi ha specificato che per donna si intende un individuo umano di sesso femminile - pensa te - e che tale vantaggio era riservato ai soli individui umani di sesso femminile, europei ed eterosessuali. La civiltà, insomma, non deve riguardare le lesbiche, le americane e le straniere in generale. Dovremmo essere civili solo tra di noi, tra pochi intimi. Che oggi vi siano problemi di intolleranza, di paura, di malcelato razzismo, di sessismo e ignoranza è cosa abbastanza ovvia.

alla ricerca di una maggiore inclusione e istruzione, più aggiornata ed efficiente, e alla sensibilizzazione delle persone. Tuttavia, mi chiedo come possiamo sperare di vincere questa battaglia se l'intolleranza, la paura, il razzismo, il sessismo e l'ignoranza provengono provengono prima di tutto dalla classe dirigente. Mi domando se un sindaco o un politico in generale debba accontentarsi di essere mera espressione delle persone che lo hanno eletto o non debba almeno cercare di essere un modello. Quel regolamento, anche se è stato cambiato e forse verrà ritirato, è stato prima pensato, scritto e presentato. Ha richiesto tempo, burocrazia e presumibilmente qualche discussione. Questo ci porta a due possibili scenari. se Carozzi credeva in quel che ha proposto, ma che ha poi cambiato o forse ritirato sotto la pressione dei *media* o di altri esponenti politici, allora siamo di fronte all'ignoranza, al razzismo e al sessismo. se Carozzi non ci credeva, allora ha agito per strizzare l'occhio alle persone che coltivano quei sentimenti per dimostrare di essere l'uomo che merita il loro voto. In tal caso, saremmo di fronte a quel populismo becero di cui la stampa a quel populismo becero di cui la stampa e i cittadini stessi ci accusano ormai da anni; lo stesso che ha contribuito a rovinare il rapporto di fiducia tra popolo e istituzioni.

Vorrei che eventi siffatti non rimanessero, come spesso accade, soltanto a beneficio della stampa, che può costruirci qualche articolo canzonatorio sopra. Vorrei che, quando un dirigente pubblico dimostra atteggiamenti razzisti e sessisti, non diventasse solo una barzelletta, ottenendo solo qualche amaro sorriso e alzata di spalle e poi domani è un'altro giorno e si vedrà. Compito dei politici è anche di proteggere la democrazia e i valori che abbiamo stabilito appartenere a questo Paese. Dovremmo chiederci, quando accantoniamo quando accantoniamo certi eventi con una scrollata di capo, se effettivamente lo stiamo facendo con la serenità e la dedizione che meritano. Come è scritto nell'ultimo libro di Luciano Violante, la democrazia non esiste in natura, è il frutto della ragione e del desiderio di libertà e, per questo, va curata. Molti hanno creduto che la democrazia non avesse bisogno di cura perché non suscettibile di deperimento, e non è così. Condivido appieno queste parole, che ci fanno riflettere su quanto sia importante essere democratici e liberi. Ciò che dovremmo riuscire a fare è continuare nell'esercizio della democrazia e riuscire a esportarla dove oggi non c'è. Signora Presidente, il giorno 13 gennaio del 2012, nella mia Regione, la Toscana, un giovane uomo di soli trent'anni, Giuseppe Girolamo, sacrificò la propria vita per salvare quella di una piccola creatura. Il giovane era imbarcato sulla nave da crociera Costa Concordia e lavorava come musicista. Questo mio intervento, a quasi cinque anni da quella tragedia e da quell'atto, vuole sollecitare ciò che fu richiesto già da tempo, e cioè il riconoscimento del gesto tramite l'assegnazione della medaglia d'oro al valor civile. Oggi, dopo quasi cinque anni da quel giorno in cui persero la vita 32 persone, a telecamere spente e telegiornali silenti, mi sento in obbligo morale di non abbassare la guardia e di insistere per il giusto riconoscimento per l'atto eroico di quel giovane uomo. Per questo ho depositato un'interrogazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al ministro Minniti, affinché si attivino veramente e non cada tutto nell'oblio. La mia si aggiunge alle molte altre interrogazioni dei colleghi. Oggi come oggi, signora Presidente, vivere del proprio estro, vivere di musica - abbiamo appena parlato di cosa è il mondo dello spettacolo - non è semplice: bisogna essere un po' sognatori e sicuramente bisogna essere determinati nel portare avanti le proprie aspirazioni, probabilmente amanti dell'invenzione e dell'estro, sicuramente innamorati della vita. Invenzione, estro e amore non mancarono a Giuseppe in quella notte drammatica e buia in cui la sua aspirazione massima si tradusse nella decisione di cambiare la salvezza di un bimbo con la propria vita, poiché Giuseppe, il musicista, non sapeva nuotare. quanto opportuno per effettuare un abbandono nave ordinato, mettendo al sicuro passeggeri ed equipaggio, e lasciava poi cadere nel vuoto le sollecitazioni della Capitaneria di Livorno a riprendere il proprio posto, Giuseppe aveva deciso in autonomia la cosa più nobile che potesse fare: sacrificarsi per salvare la vita altrui. Tenuto conto che la legge 2 gennaio 1958, n. 13, riconosce e ricompensa il valore civile per premiare atti di eccezionale coraggio, sollecito vivamente l'interessamento da parte dei Ministri interrogati. Inoltre, ricordo che esiste una petizione lanciata in rete, dove centinaia di migliaia di cittadini

Presidente, viviamo in un periodo storico così delicato, in cui la fraternità, l'altruismo, i valori della convivenza e della vita sono avvertiti come debolezze e relitti del passato i giovani crescono nella convenzione che si ottenga rispetto e riconoscimento dalla società solo se ci si dimostra sufficientemente insensibili ed egoisti. I giovani, Presidente, hanno bisogno di esempi e modelli e credo che quello di Giuseppe Girolamo sia finalmente da riconoscere e valorizzare. Vorrei rivolgere anche un ringraziamento particolare a chi, dopo tanto tempo, ha sollecitato la mia coscienza e la mia responsabilità. È facile, infatti, nel momento della più alta risonanza mediatica, interessarsi di un tema, ma è più difficile insistere a distanza di così tanto tempo. A mia volta sono stata sollecitata e, quindi, ringrazio coloro che mi hanno rimessa davanti alla mia responsabilità. Faccio appello a tutti voi e alle più alte istituzioni affinché questo riconoscimento sia veramente concesso. *(Applausi del

relativa alla situazione, nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, di una discarica che è nata male ed è cresciuta peggio.

ha già provocato danni, avendo sversato il percolato sul letto di un torrente, a valle del quale vi sono dei pozzi